signor Ministro, onorevoli colleghi, questo provvedimento, che assume la veste di decreto-legge e che già la Camera ha approvato con modifiche il 27 gennaio

dare attuazione al principio della certezza del diritto che sottende la nostra Carta costituzionale, che è un valore costituzionale. Naturalmentela semplificazione ha vari strumenti per realizzarsi

perenzione delle norme, rinvenibile solo attraverso un complesso, articolato e difficile processo di ricerca e di interpretazione. secondo luogo, semplificazione significa anche riordinare il sistema normativo, che non si può riordinare se prima non si conosce quello che vive e quello che è morto, quello che c'è e quello che non c'è. normativa debba tendere, dal punto di vista sostanziale, a consentire interventi legislativi che realizzino

e ciò sia per il mondo delle famiglie e delle imprese sia per la stessa pubblica amministrazione, frenata nella sua azione da letture contrastanti o incerte dei testi normativi che ne regolano l'attività. Questo percorso dovrà portare anche presente nel decreto-legge in esame e non invece in altri provvedimenti relativi a questa materia, l'obiettivo cioè di creare finalmente una banca pubblica gratuita degli atti normativi quanto meno dello Stato, con l'ambizione che poi tale banca pubblica comprenda anche gli atti normativi regionali e tutti quelli che costituiscono le fonti del nostro diritto.

di poterne ricordare l'attuazione completa entro questa legislatura - la creazione di un *database*, di una banca dati molto articolata e ragionata di tutti i testi normativi (prima legislativi e poi, ce lo auguriamo, anche regolamentari) che regolano la vita dei nostri cittadini. È un sistema informatico molto complesso,

realizzare, sotto un'unica bandiera, con una sola missione, il cosiddetto taglia-leggi e il progetto «Normattiva», cioè la creazione della banca pubblica della legislazione vigente

tra lo Stato e le Regioni. La Camera ha introdotto alcune modifiche proprio per puntualizzare questo aspetto. Ricordo inoltre ai colleghi che gli interventi sui sistemi informatici sono di competenza esclusiva dello Stato, come recita il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ma è bene che le Regioni vengano coinvolte e possano esprimersi, allineare

comunque coincidano con l'entrata in vigore della cosiddetta norma ghigliottina prevista nella disposizione taglia-leggi contenuta nella legge di semplificazione n. 246 del 2005, all'articolo 14, dove si prevede un processo per arrivare non solo - voglio voglio qui ricordarlo - ad abrogare leggi, ma anche a riordinare il sistema normativo raccogliendo le leggi superstiti in settori sui quali poi possono essere operati interventi più articolati ci troviamo nella fase di pulizia degli archivi, che può sembrare un passaggio banale ma che è invece molto importante, perché qualsiasi operatore del diritto, qualsiasi cittadino che vuole avvicinarsi ad una conoscenza più diretta delle fonti del diritto si trova in grande difficoltà quando trova contenute in questi archivi, cartacei o informatici che siano, una serie di disposizioni per le quali non vi è stata abrogazione espressa.

purtroppo, lo riconosciamo - soltanto con un intervento d'urgenza quale è il decreto-legge, in attesa che si utilizzino i nuovi sistemi previsti dalla normativa ordinaria che prima ricordavo.

Signora Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, lo Stato italiano produce leggi. Tante. Più di Inghilterra e Spagna messe assieme. Talmente numerose che fino a poco tempo fa non si sapeva neppure quante fossero in vigore. La stessa Cassazione ha memorizzato nella sua banca dati solo le norme più recenti. Il nuovo Ministero senza portafoglio per la semplificazione normativa, affidato a Roberto Calderoli, già l'anno scorso aveva individuato un numero incredibile di leggi operative e aveva preso provvedimenti. Il decreto-legge n. 112 del 2008 collegato alla manovra economica, insieme ad un'opera approfondita di revisione tecnica, ha determinato l'abrogazione di 7.043 norme valutate obsolete, inutili o già implicitamente abrogate, alleggerendo di molte scartoffie le imprese, con ricadute paragonabili a discreti sgravi fiscali, senza appesantire il bilancio dello Stato. Ricordo che la burocrazia pesa sulle aziende italiane per circa il 4,6 per cento del prodotto interno lordo (75 miliardi di euro). Gli accordi europei prevedono un taglio del 25 per cento degli oneri amministrativi entro il 2012 e da subito l'applicazione delle misure previste nel decreto collegato alla manovra economica ha consentito di realizzare un risparmio superiore ai 4 miliardi di euro l'anno, in settori che con le vecchie procedure sfioravano un costo di 7 miliardi. Ed eravamo solo all'inizio. Nella legislazione italiana sono infiniti gli esempi di leggi inutili o superate, che nessuno si è mai premurato di eliminare e ci sono pure norme dimenticate che potrebbero essere utili. Per scovarle le amministrazioni pubbliche si abbonano a banche dati private, con la spesa che ne consegue. Nonostante ripetuti tentativi, infatti, l'idea di creare una banca dati pubblica non è mai andata in porto. Adesso ci pensiamo noi. Con la conversione in legge del decreto n. 200 in materia di semplificazione normativa, insieme al taglio di qualcosa come 29.000 leggi, superate perché di fatto tacitamente abrogate da leggi successive o perché riferite a fatti del passato ormai privi di rilievo o perché in contrasto con i princìpi dell'ordinamento giuridico attuale, si procederà alla creazione di un archivio informatico pubblico completo della legislazione statale vigente. Una banca dati gratuita e accessibile a tutti gli utenti, perché politica e istituzioni devono essere più trasparenti e vicine ai cittadini. E si risparmia. Eccome si risparmia! Milioni di euro. Pochi sanno che la marchiatura e l'inserimento di ogni singola legge costa 2.000 euro. Se moltiplichiamo per le 29.000 norme di questo provvedimento, che vanno a sommarsi alle 7.000 della legge precedente, fanno 72 milioni di euro l'anno risparmiati, a fronte di uno stanziamento di 3,8 milioni per la banca dati normativa. Certo, in un ginepraio del genere può capitare di trovare qualche legge che merita di essere salvata, norme che di fatto è come se non esistessero, perché nessuno le conosce, delle quali non c'è traccia in nessuna banca dati e che emergono proprio grazie al lavoro del Ministero alla semplificazione. Ci sarà il tempo per recuperarle. Intanto eliminiamo le norme che regolano la pesatura dei muli alle dogane, la tassa per la bonifica dell'agro romano (datata 11 dicembre 1878, come se lì ci fossero ancora le paludi) e la legge sui piccioni viaggiatori, che disciplina l'uso dei volatili per la trasmissione a distanza. E lavoriamo a un sistema federale, agile e poco oneroso, dove gli amministratori sono caricati di responsabilità precise ed è loro interesse far funzionare la macchina dello Stato, a tutto vantaggio dei cittadini.

la natura di questo provvedimento che con gli obiettivi che si propone - la banca dati unitaria, lo *stock* legislativo ridotto, la semplificazione normativa ha per noi una valenza prevalentemente tecnica, e tale può e deve restare se non si intraprendono procedure e percorsi di volta in volta improvvisati che finirebbero per complicare la materia anziché semplificarla. fatto che la finalità di realizzare un ordinamento moderno, fondato su norme semplici, snelle, comprensibili, a beneficio dei princìpi di efficacia, efficienza, speditezza, rappresenta per noi dell'Italia dei Valori un obiettivo di buona politica, condiviso d'altronde già da tempo da tutte le altre forze politiche. Non a caso, si tratta di uno dei pochi argomenti rispetto ai quali, dal 2000 ad oggi, i vari Governi che si sono succeduti si sono mossi tutti nella stessa direzione. Per noi dell'Italia dei Valori in questo campo un valore semplice e fondamentale è quello di affermare che dietro ogni scelta legislativa, amministrativa, e quindi politica, deve esserci la vita del cittadino utente, del cittadino consumatore, di chi è amministrato e deve riconoscersi l'attività di un'impresa che deve vedere nella pubblica amministrazione uno strumento per la competitività del nostro Paese e non un ostacolo o un costo aggiuntivo. costo aggiuntivo. Considerati questi due aspetti, vogliamo mettere in evidenza alcuni rilievi tecnici e alcune distinzioni che non consideriamo comunque marginali.

Troviamo non poche difficoltà a ricercare una necessaria urgenza per portare a conclusione un programma di informatizzazione della normativa vigente avviato con l'articolo 107 della finanziaria per l'anno 2001; un intervento, quindi, iniziato con il Governo Prodi e portato avanti con il provvedimento noto come taglia-leggi, varato dal Governo di centrodestra nel 2005. all'interno di questo quadro si collocano poi due interventi successivi, quello dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 (si trattava in quel caso di 3.300 atti normativi) il decreto-legge oggi in discussione, che prevede l'abrogazione di quasi 30.000 atti emanati prima del 1947, e quindi in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. signora Presidente, signor Ministro, non è convincente quanto è stato detto sul rischio della perdita delle risorse di copertura, visto che la legge finanziaria 2008, all'articolo 2, nel recare alcune disposizioni tendenti a dare un nuovo impulso alle attività di informatizzazione, stabiliva che i fondi non impegnati negli esercizi precedenti rimanessero destinati in via prioritaria - in via prioritaria - al completamento delle attività di informatizzazione. Così come non è convincente quanto è stato detto sulla necessità, con questo nuovo decreto, di salvare ciò che deve essere salvato, visto che l'articolo 3 del questo decreto espunge 60 atti normativi di rango primario elencati nell'Allegato 2 del decreto-legge n. 112, che dovevano intendersi abrogati a decorrere dal 22 dicembre. Ciò mette in risalto un secondo elemento: la fretta molto spesso fa i gattini ciechi. Il decisionismo di questo Governo finisce spesso in propaganda nazionale. La tanto decantata rapidità di esecuzione ha significato ora e in altre occasioni che abbiamo visto rapidità di errore, per cui, per paradosso, un decreto-legge ha prodotto un altro decreto-legge. Non a caso il decreto oggi in discussione è stato emanato proprio il 22 dicembre, ossia l'ultimo dei 180 giorni in cui era possibile salvare una serie di leggi abrogate e tagliate dal decreto n. 112, in relazione alle quali ci si era resi conto di alcuni vuoti che si sarebbero prodotti. Queste ultime ragioni ci aiutano a comprendere che, se vogliamo andare realmente avanti nella direzione di superare la nostra normazione, che è sempre più obsoleta, ostica, sempre più per addetti ai lavori, il Governo deve agire non soltanto con semplici interventi *spot*, ma con un piano organico dal punto di vista dell'innovazione e della stessa semplificazione amministrativa. Per questo deve essere chiaro che il solo criterio quantitativo non basta. L'operazione dell'abrogazione delle norme è una delle più complesse e al tempo stesso soggettive. Alla base di una raccolta di norme, per accertare se sono vigenti, non c'è soltanto un elenco come quello telefonico. E quando il legislatore compie operazioni relative all'abrogazione, in diversi casi si lascia un margine di soggettività all'interpretazione. Così come, se vogliamo andare nella direzione non solo di una produzione normativa meno prolifica ma soprattutto di qualità formale e sostanziale migliore, migliore, non vi è dubbio che non basta semplificare soltanto, tagliando per il passato, senza porci da oggi il problema della semplificazione sul piano normativo, di una nuova cultura della delegificazione, dato che siamo di fronte ad un evidente, chiaro affollamento di norme e di leggi. Molto significativo è un articolo apparso tempo fa sul «Corriere della Sera», in cui si faceva un esame di quanto era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del mese di novembre: oltre 4.000 tra provvedimenti, leggi, regolamenti e quant'altro. I cittadini e le imprese sanno che l'ipertrofia normativa è un costo economico, finanziario, sociale che nessun Paese moderno può permettersi più di sostenere e sopratutto sanno che l'ipertrofia normativa è alla base della stessa incertezza del diritto. Troppe volte e troppo spesso in questo campo vi è stata una facile strumentalizzazione politica nell'accusare le disfunzioni della pubblica amministrazione e l'inefficienza dei pubblici dipendenti, senza andare alla fonte di questi problemi.

questo provvedimento un nuovo passo di un percorso che porti finalmente rimedio ad una legislazione che sia più ordinata, più consultabile, più fruibile, ma soprattutto più vicina al cittadino.

Come poteva permanere una situazione del genere, una giungla normativa complessa, che forse nessuno conosceva fino in fondo?

esaminato dalla Camera dei deputati; sono state apportate delle modificazioni, è stato migliorato il testo ed è stato fissato il termine del 16 dicembre 2009 per segnalare, se ve ne fossero, abrogazioni inopportune. Mi sono chiesto per quale motivo un lavoro del genere non fosse mai stato fatto prima o, perlomeno, non avesse trovato una sua compiutezza. Ho cercato di darmi delle risposte. Costituire una vera e propria banca dati della normativa statale vigente si è dimostrato negli anni un obiettivo estremamente più complesso di quanto era stato ipotizzato in origine. Ciò era dovuto essenzialmente a tre ordini di motivi.

e una non omogeneità delle norme sulle fonti, sia di produzione sia di conoscenza, nel medesimo periodo. In secondo luogo, la frammentazione e il disordine dell'ordinamento, dovuti anche alla scarsa importanza tradizionalmente attribuita dal legislatore alla qualità della legislazione, con la conseguente difficoltà di identificare la normativa vigente anche in relazione alle la povertà del patrimonio di raccolte elettroniche oltre alla mancanza di una raccolta completa degli atti normativi, che si registrano anche per i sistemi generalmente ritenuti più affidabili. Detto questo, che in parte tranquillizza la coscienza, ho sentito che qualcuno ha voluto liquidare il provvedimento in esame come una norma tecnica, una norma senza veste politica, politica, che cerca cioè di trovare una soluzione tecnica ad un problema reale. Al contrario, credo che suo valore politico sia alto, molto alto, perché secondo noi della Lega Nord Padania la trasparenza, la semplicità, la facile accessibilità alle norme vigenti in questo Stato sono uno dei tanti pilastri fondanti della democrazia. C'è voluto un Ministro della Lega per concretizzare tale obiettivo e noi tutti della Lega Nord Padania gliene siamo grati.

Voglio porre l'accento sulla sostanza di questo provvedimento, non solo formale ma anche di buona politica, che ha permesso una convergenza sui metodi di intervento del Parlamento rispetto al decreto-legge in discussione. Ad esempio, il controllo delle disposizioni che dovranno essere abrogate dovrà essere il più possibile accurato, assicurando una diffusa verifica di esse da parte di tutti i soggetti in grado di fornire un contributo volto ad accertare l'eventuale necessità di sopravvivenza della normativa ritenuta indispensabile.

Signora Presidente, credo che il provvedimento che stiamo discutendo debba avere un valore di stimolo sia per noi parlamentari, nel cominciare ad immaginare un lavoro legislativo di maggior qualità, sia per le altre entità legislative quali le Regioni, per non gravare i cittadini con un eccesso di norme. Esso deve rappresentare altresì un momento che ci induca, come Parlamento, ad accelerare l'azione volta a rendere omogenea la legislazione per materia, muovendoci in fretta verso l'importante traguardo dei testi unici. Senza enfasi, come quella data a volte ad altri provvedimenti, ritengo che stiamo comunque varando una riforma, un atto dovuto ai cittadini, un passaggio importante verso una trasparenza che deve essere uno dei mezzi per avvicinare i nostri concittadini alle istituzioni e un modo per rendere più credibile anche chi, come noi, nelle istituzioni lavora. dal mio punto di vista, non stiamo realizzando solamente un atto di buona amministrazione: stiamo facendo buona politica.

e quindi ha una storia che è profondamente radicata nella cultura di governo a cui io mi sento di appartenere. Semmai ci sarebbe da chiedersi i motivi per cui abbiamo dovuto aspettare fino al 2005 prima di arrivare ad una legge delega che mettesse in atto quel percorso che poi ci ha permesso, nel 2007, di arrivare alla prima relazione

abbiamo avuto altre testimonianze all'inizio di questa legislatura, in cui arrivano in Aula provvedimenti la cui storia nasce

quello dell'informatizzazione, e quindi della facilità di accesso e di consultazione, e quello della semplificazione. Già i colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto hanno sottolineato

in questo campo è cattiva consigliera. L'episodio più noto che voglio citare è quello delle tariffe delle Ferrovie dello Stato, ma ci sono state anche altre sviste,

l'ordine del giorno fatto proprio anche dalla 1a Commissione, che credo troverà totale recepimento in quest'Aula, ci permettono almeno di mitigare

Mi riferisco all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la cosiddetta taglia-leggi, che prevede tre passaggi fondamentali. Innanzitutto, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge il Governo è chiamato a individuare disposizioni legislative

Si prevede, inoltre, che entro i successivi 24 mesi il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970,

l'abrogazione automatica delle disposizioni legislative. Si tratta, quindi, di un percorso in qualche misura incrociato ma anche inverso a quello che stiamo seguendo.

con uno strumento appropriato, quello della delega legislativa, con un coinvolgimento parlamentare. Questa coniugazione ottimale non è però attribuibile alla decretazione d'urgenza

quale lavoro ci aspettiamo svolga il Governo per investirne successivamente il Parlamento. L'altro elemento di problematicità, come avevo già anticipato, è che questo decreto va a sanare gli errori

settimana licenzierà una relazione senz'altro tardiva rispetto ai tempi della legge, ma comunque tempestiva per quanto riguarda il succedersi delle legislature, il cambiamento dei Governi, l'entrata in funzione della Commissione e, soprattutto,

prevede una fase abrogativa, ma anche una fase e una funzione di un riordino della normativa che viene assunta come vigente; quindi ha questo doppio contenuto che, ripeto, sta impegnando gli uffici del Governo

anche una serie di norme a regime sulla chiarezza dei testi, sui regolamenti, sui Testi unici compilativi, che dovrebbero aiutare - spero che il Governo ne faccia tesoro e le utilizzi - un percorso di legislazione e comunque di normazione ordinata e razionale, sulla quale poi innestare di volta in volta gli interventi del legislatore nazionale. Questo può essere un obiettivo utopico, ma ritengo che sia nostra responsabilità farcene carico. Sottolineo che la presenza di un Ministro *ad hoc* per questa missione testimonia l'attenzione, confermata da parte del Governo Berlusconi, su questo progetto. Il decreto-legge in esame

aspiriamo allo zero per cento, ma come primo esperimento in questo campo, considerata la delicatezza e la complessità della materia, mi sembra che sia una prova riuscita, con correttivi successivi, tra i quali questo decreto-legge. con tutto il processo di semplificazione che è funzionale alla creazione dell'archivio, come la creazione dell'archivio è funzionale ad un processo di chiarezza legislativa. Le due cose stanno insieme. unificata la missione in capo ad un unico Ministro, vengono unificate le risorse, viene unificata l'organizzazione e vengono unificate anche le logiche, senza disperdere il patrimonio che finora finora abbiamo accumulato, grazie al lavoro svolto in questi anni attraverso il legislatore, ancorché di diversa colorazione politica. Ripeto, questo è un passaggio significativo; ci saranno altri passaggi. Ci auguriamo (e presentiamo un ordine del giorno in materia firmato da me) che non si ricorra più al decreto‑legge, perché ora siamo

del decreto legislativo.

Per me 120 miliardi di lire sono un ottimo motivo di necessità e urgenza e, soprattutto in periodi di crisi, cerchiamo di usarli meglio ed evitare di buttarli via.

centinaia di migliaia di posti di lavoro e fa tirare la cinghia a milioni di famiglie, la RAI, finanziata dal canone dei cittadini, si permette di elargire un milione di euro a Paolo Bonolis per Sanremo che, tra l'altro, di fronte alle critiche, ha definito infelici quei parlamentari che hanno ritenuto scandalosi quei compensi. Il quotidiano «La Stampa» del 15 febbraio ha commentato come affari di famiglia gli appalti del Festival di Sanremo, affidati alla scuderia di Lucio Presta, l'agente di Bonolis, che vede in campo il suo *staff*, dal direttore d'orchestra al direttore artistico, dagli autori come Lanza e Salvati alla - ciliegina sulla torta torta - signora Sonia Bruganelli, ovvero la moglie di Paolo Bonolis, che si sta occupando del *casting*, o meglio «solo di alcuni momenti del Festival» - sottolineano fonti RAI -«e cioè delle modelle, dei ragazzi...». Insomma, la famiglia è al completo, non solo per Bonolis, ma anche per Presta che oltre al *cast* - per così dire tecnico «scaricherà» sul palco dell'Ariston una serie di personaggi legati al suo ruolo. Insomma, il vero *deus ex machina* degli artisti non sembrerebbe tanto la RAI, che pure finanzia la gara canora, quanto il manager delle *star*. È lui, infatti, che tratta i compensi dei *big* principali, che rilancia sui diritti di Benigni e che, forse casualmente, sceglie e trova le migliori risorse per Sanremo proprio nel guardaroba di casa, nel cosiddetto *book* di famiglia. Esistono poi rapporti pregressi tra Lucio Presta ed il direttore di Raiuno Fabrizio Del Noce, sui quali occorre fare chiarezza. Signora Presidente, siccome sono tra quei tra quei parlamentari infelici che hanno presentato interrogazioni al riguardo, chiedo che il Ministro dell'economia e delle finanze o quello dello sviluppo economico vengano a rispondere su questi scandalosi compensi, ma anche sulla violazione degli obblighi di legge, previsti dall'articolo 3, comma 44, della legge